ogni venti minuti nel mondo una persona, spesso una bambina o un bambino, muore o viene mutilata da una mina antipersona. Sono passati dieci anni dal 1° marzo 1999, data in cui è entrato in vigore lo storico Trattato di Ottawa per la messa al bando delle mine antiuomo. Il Trattato è stato adottato con la firma di 122 Stati, che si erano impegnati ad impedire ogni produzione, uso, stoccaggio ed esportazione di mine antipersona, a distruggere entro quattro anni tutte le mine antipersona esistenti nei rispettivi arsenali, a bonificare le aree minate nei proprio territorio entro dieci anni, a fornire assistenza tecnica e finanziaria per le operazioni di sminamento e assistenza alle vittime. L'Italia ha firmato il Trattato di messa al bando delle mine il 3 dicembre 1997, ed è diventata Stato parte del Trattato il 1° ottobre 1999. Dal 1995 il Parlamento italiano interagisce costantemente con la campagna italiana contro le mine per definire una legislazione nazionale volta al bando totale di questi ordigni. Con la legge 7 marzo 2001, n. 58, è stato istituito il Fondo per lo sminamento umanitario, assistenza alle vittime e sensibilizzazione delle popolazioni civili. Ora il numero degli Stati aderenti al Trattato ha raggiunto quota 156. Solo 39 sono i Paesi che non hanno ancora aderito, tra cui potenze mondiali quali gli Stati Uniti, la Cina, l'India, la Russia ed il Pakistan. Noi oggi qui crediamo che il dovere di chi ricopre un ruolo di rappresentanza nelle istituzioni, a partire dal Senato, sia non solo e non tanto quello di celebrare con le parole un avvenimento così significativo, ma soprattutto di rendere coerente e concreta l'adesione che il nostro Paese ha dato a quel Trattato ormai molti anni fa. Dal 30 novembre al 4 dicembre di quest'anno, a Cartagena in Colombia, avrà luogo la seconda importante conferenza di revisione della Convenzione. In preparazione di questa Assemblea, il 4 aprile scorso, si è celebrata la quarta giornata internazionale per la sensibilizzazione sul problema delle mine e sul sostegno alla *mine action* delle Nazioni Unite. A Roma è venuta la cambogiana Song Kosal, ambasciatrice per i giovani della campagna internazionale per la messa al bando delle mine, rimasta vittima di una mina all'età di sei anni. Song Kosal, oggi ventiquattrenne, saltò su una mina mentre lavorava nelle risaie e raccoglieva legna per il fuoco. Nessuno sospettava che in quel campo ci fossero delle mine. Ha sofferto all'inizio del suo calvario 1'emarginazione di quanti risultano menomati nel corpo e quindi spesso emarginati nei loro Paesi e relegati, tanto più se donne, a ruoli subalterni. Ora Song gira il mondo a portare la sua testimonianza e si è rivolta alle autorità italiane perché massima fosse la sensibilizzazione sul problema delle mine e a sostegno della *mine action*. «L'Italia ci deve ascoltare» - ha dichiarato - «Servono ancora fondi per la bonifica di terreni minati e per l'assistenza e la reintegrazione socioeconomica delle vittime di mine e ordigni inesplosi». Il 1° aprile Song Kosal ha incontrato Sua Santità Benedetto XVI e non è secondario ricordare che il Papa all'*Angelus* del 5 aprile è autorevolmente intervenuto, non solo per accentrare l'attenzione sulla Giornata internazionale indetta dall'ONU, ma anche per ricordare la necessità della rapida entrata in vigore della Convenzione di Oslo per la messa al bando delle bombe a grappolo. Essa ancora deve essere ratificata dal nostro Paese, uno dei primi firmatari. Il sostegno del Papa è andato anche a «garantire» - sono le sue parole - «la necessaria assistenza alle vittime di tali armi devastanti». Oggi infatti, sono ancora decine di migliaia le mine, molte delle quali anche di produzione italiana, disseminate in quasi tutti i Paesi che hanno una guerra in corso o che sono usciti da conflitti armati. I maggiori Paesi detentori di mine sono: la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, la Corea del Nord, la Corea del Sud, l'India, I numeri del disastro riferiscono di centinaia di migliaia di vittime nel mondo, di più di 80 Paesi in via di sviluppo con presenza di mine sul territorio, di 200 milioni di mine depositate negli arsenali militari (una mina ogni 48 abitanti del pianeta e una per ogni 16 bambini).

I processi di sviluppo e di costruzione rischiano di non poter mai iniziare perché è indispensabile che si realizzi preventivamente la bonifica del territorio e delle infrastrutture. Nell'attività di sminamento resta centrale il problema della localizzazione degli ordigni, ma esiste anche quello della loro eventuale mobilità. Infatti, non di rado accade, come nel Laos che è un Paese gravemente infestato, che, quando si abbattono consistenti piogge monsoniche, piogge monsoniche, gli ordigni si disincaglino dal suolo per venire dislocati altrove insieme a detriti fangosi formati da ruscelli temporanei. Per consentire nuovamente alla popolazione di riappropriarsi di campi coltivabili, di canali per l'irrigazione, di strade dell'uso di importanti testimonianze archeologiche e, quindi, di attrazioni turistiche utili allo sviluppo del Paese, spesso sarebbe sufficiente una adeguata dotazione tecnica, a partire dai *metal detector*. Un'esperienza d'eccellenza che voglio ricordare è quella che si realizza in Laos,

Non diversa e quindi aggiuntiva è la drammatica situazione conseguente alla presenza di bombe a grappolo nel territorio. Tutti sanno cosa sono le *cluster bombs*: armi di grandi dimensioni, usate per la prima volta nella seconda guerra mondiale, lanciate dagli aerei o dai sistemi di artiglieria, che si aprono a mezz'aria spargendo ad ampio raggio centinaia di submunizioni più piccole. Le submunizioni sono progettate per esplodere al momento dell'impatto con il suolo, ma se non esplodono, per i motivi più vari - e questo succede spesso, tanto che si parla della possibilità di non esplosione che va dal 5 al 20 per cento - allora restano nel terreno come le mine antipersona, uccidendo e menomando chiunque le tocchi.

E' vero che l'Italia rispetto alle *cluster bombs* può dire di essere un Paese nel quale ormai non si producono più tali ordigni, anche se la Simmel Difesa S.p.A, ex azienda italiana che nel marzo 2007 ha ceduto l'intero capitale

Per quanto riguarda i danni dalle mine *cluster,* voglio qui ricordare che le menomazioni prodotte evidentemente non feriscono solo il corpo, ma profondamente anche lo spirito, se è vero quello che è stato recentemente riferito da un professore associato dell'università di Kabul, cioè che il 65 per cento degli uomini che scelgono di uccidersi seminando morte, gli uomini bomba che portano altro terrore nei luoghi di guerra, risulta essere stato precedentemente ferito e menomato. Il Senato ha già preso posizione il 28 maggio dello scorso anno votando una mozione unitaria con la quale impegnava il Governo ad assumere nell'ambito della Conferenza di Dublino, preparatoria per Oslo, e nel rispetto degli impegni internazionali delle operazioni di pace, una posizione decisa per la messa al bando delle bombe a grappolo. Voglio ora esprimere la mia soddisfazione perché oggi qui siamo riusciti a trovare una soluzione condivisa. Parlo di un ordine del giorno a firma Contini, Amati, Torri, Caforio, Fosson: sono i primi firmatari delle mozioni depositate che, quindi, evidentemente, ritireremo, perché abbiamo questo ordine del giorno condiviso e già depositato.

ad adoperarsi per reperire risorse in favore dello sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58; a ratificare in tempi brevi il Trattato di Oslo, permettendo all'Italia così di essere tra i primi 30 Paesi, che consentiranno l'entrata in vigore del Trattato medesimo;

Questo risultato mi sembra particolarmente importante in sé. Voglio inoltre ricordare che su questo tema numerosi sono stati in questi giorni gli enti locali (Comuni, Province e Regioni) che hanno inteso far pervenire analoga richiesta di impegno al nostro Governo, con mozioni e ordini del giorno assai spesso unitari. Hanno già votato in questo senso ordini del giorno e mozioni i Consigli regionali del Piemonte, della Toscana, delle Marche, del Lazio; Consigli provinciali di Bologna, Ancona, Novara, Roma, Macerata, Ferrara e Vibo Valentia e tanti Consigli comunali, tra cui Avellino, Perugia, Senigallia, Lioni,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori vorrei esprimere pochi e semplici concetti per motivare il valore e il peso dell'ordine del giorno di cui discutiamo oggi. Infatti, il Gruppo dell'Italia dei Valori intende porre l'accento sull'importanza che gli accordi internazionali già raggiunti, e quelli che si raggiungeranno, perseguano efficacemente gli obiettivi che si prefiggono. Secondo quanto stabilito nelle Convenzioni di Oslo e Ottawa, l'Italia si impegna a procedere alla distruzione di tutti gli *stock* di mine antipersona e *cluster bomb* e ne vieta inoltre la produzione e il commercio. Sono convinto che ciascuno dei colleghi qui in Aula oggi ha ben presente l'enormità e la gravità dell'impatto umanitario causato dalle esplosioni di mine antipersona, che provocano un alto numero di incidenti mortali e le cui vittime sono rappresentate per il 98 per (cioè la quasi totalità, colleghi!) da civili, tra cui molti bambini. Per avere anche solo un'idea delle proporzioni enormi di questa piaga basti pensare all'esempio del Libano: diverse organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU, stimano che solo in Libano vi siano almeno 100.000 ordigni inesplosi. Colleghi, proprio in Libano i nostri soldati sono, ormai da tempo, impegnati in una missione tra le più importanti e delicate per le relazioni internazionali del nostro Paese, missione che peraltro guidiamo dal 2007.

civile che consegue all'utilizzo di questo tipo d'arma e che quindi rappresenta un grosso ostacolo allo sviluppo di quei Paesi coinvolti nei più recenti conflitti internazionali. Infatti, per gli Stati aderenti alle convenzioni prima citate, è previsto anche l'impegno a svolgere azioni di assistenza alle vittime, non riferendosi esclusivamente agli individui sopravvissuti all'esplosione di questi ordigni, ma comprendendo anche le loro famiglie e le comunità di appartenenza, compreso il loro reinserimento socioeconomico, la prevenzione dal rischio per le popolazioni dei territori interessati, l'attuazione di programmi di bonifica umanitaria. Proprio per la realizzazione di questi obiettivi, con la legge 7 marzo 2001, n. 58, l'Italia ha istituito il Fondo per lo sminamento umanitario, completamente in linea con i parametri delle suddette convenzioni. Eppure, contravvenendo alle dichiarazioni di Oslo, il Governo italiano ha prima dimezzato (nell'ambito della legge finanziaria per il 2004) e poi azzerato il Fondo per lo sminamento umanitario, non riconfermando il suo impegno nella *mine* *action* e nell'assistenza alle vittime. azzerato il finanziamento destinato al Fondo per lo sminamento umanitario, come può il nostro Paese presentarsi ai futuri importanti appuntamenti internazionali senza essere accusato d'aver ridotto il proprio impegno nella lotta contro la piaga delle mine antipersona? Ciò non renderebbe certo onore a un Paese ex produttore ed esportatore, che ha fatto del rispetto dei diritti umani la sua bandiera. Da qui l'esigenza avvertita dall'Italia dei Valori di ritirare la mozione che portava la firma mia e dei miei colleghi e contestualmente di sottoscrivere l'ordine del giorno a firma della senatrice senatrice Contini, unanimemente con tutti i rappresentanti dei Gruppi all'interno della Commissione difesa. L'ordine del giorno è valutato con soddisfazione dal mio Gruppo, in quanto esprime comunque volontà di impegnare il Governo al reperimento dei fondi utili a rifinanziare urgentemente il Fondo per lo sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, permettendo così di assolvere agli impegni presi e porre in essere tutte le azioni politico-diplomatiche atte a garantire il necessario appoggio finanziario per continuare a sostenere tutte tutte le attività dirette a conseguire l'obiettivo di liberare l'umanità dal terrore delle mine antipersona e dai residui inesplosi delle bombe a grappolo, contribuendo a costruire un mondo più sicuro per le generazioni presenti e future.

esteri*. Signor Presidente, cari colleghi, il Governo prende atto con viva soddisfazione del lavoro che è stato fatto dai vari Gruppi parlamentari per arrivare ad un unico ordine del giorno

Il Fondo è nato per sostenere le attività di bonifica e di prevenzione ed è stato costituito nel 2001; è stato il segnale più visibile dell'impegno del Governo italiano in materia. l'Italia è stata uno dei primi Paesi ad eliminare dai propri magazzini qualunque mina e a non produrne più, pur

Il Fondo che gestisce il Ministero degli affari esteri agisce secondo linee guida che rispondono alla Convenzione di Ottawa e alle logiche degli impegni sottoscritti alla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, che in questo senso vengono analogamente considerate come le mine antipersona. Le risorse vengono impiegate sulla base di criteri di priorità umanitaria l'utilizzo di questo Fondo è preceduto sempre da una consultazione con le organizzazioni non governative attive in tale settore e che fanno parte del Comitato nazionale per lo sminamento umanitario.

serve invece a finanziare le organizzazioni non governative che a questo si dedicano. Il Governo vuole sottolineare che questo Fondo è finanziato dal Governo, che la stessa legge n. 58 del 2001 prevede contributi e donazioni concesse da privati, enti o da organizzazioni.

Tale progetto, con un'iniziativa finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'azione umanitaria, è già stato presentato alle organizzazioni e ha già avuto il consenso della Croce Rossa e di alcune delle più importanti ONG che operano in questo campo.

parlamentari qualche volta sono molto lunghi. Comunque, ripeto che il Governo accetta questo impegno così com'è e ovviamente è d'accordo a svolgere un'azione politica atta a sollecitare in tutti i luoghi della diplomazia internazionale, delle istituzioni europee e dell'ONU, i Paesi che non hanno ancora sottoscritto i Trattati di Ottawa e di Oslo, peraltro, come ha evidenziato la senatrice Amati, che molti sono i firmatari ma che i non firmatari sono alcuni dei Paesi più importanti, dagli Stati Uniti, all'India alla Cina. Comunque l'impegno italiano non verrà certamente meno.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, esprimo con pochi concetti il voto favorevole del mio Gruppo alla mozione avente come prima firmataria la senatrice Amati. Le mine antiuomo sono state oggetto di un lungo dibattito etico a livello internazionale a causa del pericolo che rappresentano per i civili anche dopo la fine del conflitto in cui vengono impiegate. Un esempio tipico sono le cosiddette mine farfalla, usate dall'esercito sovietico in Afghanistan, che hanno un curioso aspetto e sembrano, paradossalmente, simili a giocattoli.

Un effetto simile a quello delle mine antiuomo è inoltre generato dalle cosiddette bombe a frammentazione, che vengono fatte esplodere in aria prima che impattino con il suolo, creando delle schegge che mantengono il loro carico esplosivo per anni. anni. Cito solo qualche esempio sugli effetti dell'uso delle mine terrestri. Per sminare l'Afghanistan, agli attuali ritmi, occorrerebbero circa 4300 anni. Un'indagine realizzata in Afghanistan sui feriti delle mine antiuomo chiarisce che la maggioranza delle vittime delle mine sono civili. Solo il 13 per cento dei feriti era costituito da militari; le vittime delle mine sono state colpite per l'8 per cento durante il gioco,

Oggi, quindi, sono i civili a pagare per la guerra. Nella Prima guerra mondiale, all'inizio del secolo, i civili rappresentavano solo il 15 per cento delle vittime. Come si può notare, la situazione di oggi si è capovolta rispetto all'inizio del secolo e per questo la guerra moderna è diventata molto più disumana e ripugnante perché a farne le spese sono gli innocenti. Il Trattato di Ottawa e la più recente Convenzione di Oslo si completano reciprocamente avendo come obiettivo la salvaguardia delle popolazioni civili in tempo di conflitto e post-conflitto e la distruzione delle mine antiuomo.

teatro di guerre e di poter sostenere le persone disabili, vittime delle mine antipersona.

da svariati anni, tant'è vero che nessun Governo, sia di centrodestra sia di centrosinistra, si è mai sottratto a questa volontà.

È anche il caso di ricordare che tra le zone maggiormente colpite ed infestate da questi ordigni c'è l'Afghanistan, dove

è quella giusta. Siamo congiuntamente convinti che l'operazione che stiamo facendo sia di massimo livello e chiediamo quindi con convinzione una ripresa dell'impegno da parte del nostro Paese su questo tema in maniera determinata e seria.

Lo sminamento umanitario è una parte importante di un percorso di redenzione di quegli ambienti sconvolti dalla guerra, ma molto lunga resta purtroppo la strada da percorrere. Mi corre un pensiero di logicità. Forse è così perché l'ambizione di coloro che hanno sostenuto la campagna contro le mine antipersona è quella di umanizzare tale attività

lo dichiariamo con un sentimento umanitario e, soprattutto, auspichiamo che ci sia un profondo convincimento morale

Gli illustratori potranno intervenire per 10 minuti ciascuno. Ha facoltà di parlare il senatore Gallo per illustrare la mozione n. 57.

Signor Presidente, illustri rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, la mozione n. 57 è stata presentata il 6 novembre 2008. Alla mia firma e a quella del senatore Izzo si sono aggiunte quelle di altri 86 senatori, per un totale di 88 firme, tutti senatori del PdL, di tutte le Regioni d'Italia. Ciò significa che molti parlamentari hanno sottoscritto l'iniziativa, a dimostrazione del fatto che la mozione in esame non rappresenta una rivendicazione territoriale né tanto meno un contributo assistenziale in favore delle Regioni del Sud, ma propone la realizzazione di un'infrastruttura strategica che riduce drasticamente il *gap* infrastrutturale del Sud, specie dopo un anno di polemiche in merito all'utilizzazione dei fondi FAS. Quali sono i fatti su cui poggia la mozione? Il 18 dicembre 2001 (era al Governo Silvio Berlusconi), il Presidente del Consiglio, il Ministro delle infrastrutture e il Presidente della Regione Campania hanno sottoscritto l'Intesa generale quadro con la quale veniva condiviso il Programma di infrastrutturazione dell'intero sistema della mobilità e della logistica regionale. Il 21 dicembre 2001 il CIPE, con delibera n. 121, recepiva in particolare il contenuto della predetta Intesa, inserendo il Programma della stessa nel quadro degli interventi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Detta Intesa generale quadro individuava otto distinte aree riguardanti opere di preminente interesse nazionale. Tra queste, l'area n. 1 (Corridoi ferroviari: completamento del sistema Alta velocità/Alta capacità e sua integrazione con il sistema ferroviario regionale) prevede, tra l'altro, in particolare, l'opportunità di avviare a realizzazione l'evoluzione verso Sud e verso Est del sistema Alta velocità/Alta capacità attraverso il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Napoli-Foggia-Bari.

l'impegno di inserire tra gli interventi della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (la cosiddetta legge obiettivo) il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari con le caratteristiche di linea ad Alta capacità. Ritenuto che nell'ambito di tutti i sopra citati impegni assunti dal Governo sarebbe opportuno inserire (ed è questo il senso della mozione, anche in aggiunta alla priorità da dare alla linea Napoli-Bari) linea Napoli-Bari) il prolungamento delle opere infrastrutturali fino alla Provincia di Lecce, onde evitare che il Salento rimanga l'unica area della Regione priva di collegamenti moderni ed efficienti con il resto Paese, è nata la mozione che impegna il Governo

di generare nuova economia e nuovo rilancio dell'economia. Questa considerazione era stata sollevata con la mozione sottoscritta da tanti senatori per poter essere

La dorsale adriatica da Foggia a Lecce rappresenta la parte terminale del Corridoio 8 che, attraverso l'asse Bari-Napoli, si collega al Corridoio 1, formando un sistema di trasporti proiettato verso i Paesi dell'Est europeo.

per il paesaggio, per le sue incantevoli masserie, per il suo mare cristallino e per le sue splendide coste, ma anche per lo sviluppo di settori industriali quali l'agroalimentare, il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero. merito ai tempi, proprio venerdì scorso a Benevento il ministro Matteoli, il sottosegretario Viespoli e i Presidenti delle Regioni Puglia e Campania hanno preso parte ad una tavola rotonda in cui veniva presentato il progetto preliminare della Napoli-Bari

sufficiente ad aprire una prima *tranche* di lavori. Prende così corpo la realizzazione di questa importante arteria. Credo davvero che siamo sulla strada buona e, soprattutto, che un'ulteriore spinta verrà da questa mozione con la quale chiediamo e continueremo a chiedere il finanziamento dell'intera opera. Per quanto riguarda i vantaggi, parliamo di risparmi in ordine di tempo, di maggiore qualità, di offerte. Faccio solo qualche esempio. Roma sarà raggiungibile da Bari in sole tre ore da Lecce in quattro ore, con un risparmio di un'ora e mezzo; Napoli, sempre da Bari, sarà raggiungibile in meno di due ore, con un risparmio di un'ora e 40 minuti. Oltretutto avremo un collegamento Napoli-Bari-Lecce diretto, mentre oggi bisogna fare il cambio a Caserta, cosa del tutto assurda nel terzo millennio. Il potenziamento consentirà un aumento di 15.000 passeggeri, per un totale di 20.000 all'anno, e di 6.000 tonnellate di merci trasportate al giorno. Si prevedono impatti positivi anche sulla sostenibilità ambientale: quasi 89.000 tonnellate all'anno in meno di emissioni di anidride carbonica e 306 tonnellate in meno all'anno di emissioni di ossido di azoto. In conclusione, realizzare l'Alta velocità sulla tratta Napoli-Benevento-Foggia-Bari-Lecce significa realizzare un'infrastruttura strategica che riduce drasticamente il *gap* infrastrutturale del Sud, specie dopo un anno di polemiche - ritorno a dire - per l'utilizzazione dei fondi FAS. Grazie a quest'opera si collegheranno tra loro il Corridoio europeo 1 Berlino-Palermo con il Corridoio 8 Bari-Parma e, dunque, la dorsale adriatica con quella tirrenica. I porti di Napoli e di Bari saranno in grado di svolgere al meglio un ruolo strategico nella piattaforma logistica del Sud Europa. Il triangolo Roma-Napoli-Bari diventerà uno dei sistemi metropolitani più grandi d'Europa e con la sua rete di servizi accelererà ogni forma di scambio commerciale, culturale e turistico. Il rilancio delle infrastrutture lo abbiamo sempre detto in quest'Aula - è alla base del rilancio dell'economia e in questa situazione ha un valore doppio: da un lato, è in armonia con la direzione di marcia che il Governo sta imprimendo per superare la crisi nella quale siamo attanagliati; dall'altro, il Mezzogiorno ha bisogno di questa infrastruttura per un discorso di crescita, con un forte indotto occupazionale.

da una competizione sana fra le Regioni, da una classe dirigente capace di amministrare che vuole misurarsi sulle sue capacità e viene giudicata per quello che produce, da un'amministrazione sana che deve portare i conti a posto. posto. In questa rivoluzione culturale, quindi, una classe nuova ha bisogno di servizi che siano paritari. Quindi, i servizi devono essere comuni su tutto il territorio anche in termini di livello qualitativo.

la nostra mozione è stata animata dalla volontà di offrire non già una ipotesi necessariamente alternativa od oppositiva a quella presentata testé dal senatore Gallo, bensì di proporne una in grado di offrire davvero una visione più ampia, su cui poter far convergere indistintamente i voti dell'Assemblea e su cui impegnare davvero il Governo rispetto alle priorità infrastrutturali delineabili nel Mezzogiorno del Paese. Infatti, con il massimo rispetto per il senatore Gallo, di cui siamo soliti apprezzare il lodevole attivismo da cui è animato, a noi sembra piuttosto che la mozione voglia costituire essenzialmente l'occasione per cogliere un treno che sta partendo: la realizzazione dell'Alta capacità Napoli-Bari al fine di inserirci il prolungamento verso Lecce, giustificandolo, a nostro avviso invero un po' debolmente, come opportuno, semplicemente e soltanto opportuno. Insomma, un'opportunità tra le tante. Non viene aggiunto altro se non la preoccupazione in ultimo circa la necessità di vigilare affinché le ferrovie non riducano i servizi da Lecce verso Napoli e Roma, che sembra essere, questo sì, il vero obiettivo della mozione. Come del resto, devo dire, analogo proponimento è rappresentato dalla mozione della Lega che, per converso, richiama in opposizione alla mozione Gallo la necessità del prolungamento della TAV da Milano sino a Venezia e Trieste. Venezia e Trieste. Queste due mozioni sono la plastica rappresentazione di un quadro del Paese che la maggioranza, suo malgrado, non riesce più a comprendere e tenere unito, votando - come probabilmente magari vedremo - una mozione ed il suo contrario, rendendo quindi forse inutile anche il dibattito e le sue deliberazioni. A noi pare invece che l'occasione di parlare delle infrastrutture e dei servizi necessari nel Sud del Paese costituisse un'occasione che purtroppo capita di rado nelle Aule parlamentari e che questa, sì, fosse una occasione da non disperdere. Altro allora doveva essere a nostro avviso l'impostazione ed il taglio da dare alla discussione; un profilo che noi riteniamo più conforme a quello delle mozioni presentate dall'UDC e dall'Italia dei Valori. Valori. Con questa mozione abbiamo voluto prendere sul serio tale opportunità confidando nella possibilità di un reciproco atteggiamento di rispetto e di ascolto. Ci proponiamo pertanto di rappresentare con questa mozione il semplice, si fa per dire, stato dell'arte delle infrastrutture nel Sud del Paese e, in conseguenza delle risorse effettivamente disponibili, determinare un quadro delle priorità indispensabili. Del resto, in un momento di crisi come quello attuale, non possiamo non essere unanimemente convinti che occorra concentrare le risorse e scegliere le priorità su cui investire. Per noi e non da oggi il Sud costituisce la principale sfida infrastrutturale, non solo per il nostro Paese, ma per l'intera Unione europea se è vero, com'è vero, che la prospettiva comunitaria di sviluppo economico e sociale dell'Unione europea guarda sempre più verso il Mediterraneo e segnatamente verso la sponda Sud, e sempre più verso Est, europeo ed extraeuropeo. Pensiamo pertanto che non si debba prescindere dall'inquadramento del nostro Paese nell'ambito dei corridori paneuropei e segnatamente per il Sud di quelli costituiti dai Corridoi 1 e 8. Ed è invece proprio nel Sud del Paese che sono più vistose e stridenti le contraddizioni costituite dalle affermazioni e dagli annunci del Governo, che sembrano ricomprendere nella fantomatica costruzione del ponte sullo Stretto o nella realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria le opere onnicomprensive di una realtà invece molto più complessa ed articolata. Anche per questo il nostro Gruppo ha invece voluto presentare, come dicevo, un documento che desse nella sua interezza una visione di insieme della situazione infrastrutturale del Mezzogiorno italiano, ponendo l'accento in particolare su quelle opere senza il cui completamento non sarebbe possibile procedere al completamento dei corridoi europei. In questo senso stiamo parlando di un piano delle opere essenziali per l'infrastrutturazione necessaria del Mezzogiorno che avrebbe un costo di circa 24 miliardi se avesse in cima alla lista delle spese da effettuare almeno le seguenti voci. In Calabria, innanzi tutto, il completamento del segmento autostradale Salerno-Reggio Calabria per cui sono necessari 2,7 miliardi di euro: ad oggi la disponibilità finanziaria ammonta invece a circa 600 milioni di euro. Pertanto, colleghi della maggioranza, non è vero, come è stato sostenuto ripetutamente dal Governo, che l'opera è interamente finanziata e sarà ultimata entro il 2013. Purtroppo, la triste verità è che la Salerno-Reggio Calabria è destinata a rimanere una storia infinita e non finita di questo Paese, anche al netto dei preoccupanti stati di avanzamento lavori che si registrano. Ripeto: 2,7 miliardi di euro, e mancano ancora 2 miliardi In Sicilia l'itinerario ferroviario Messina-Palermo, che comprende il raddoppio della tratta Patti-Castelbuono: 3.950 milioni di euro (circa 4 miliardi),

di euro. Il ponte sullo Stretto costa invece 6 miliardi di euro, di cui soltanto 1,3 attualmente di provenienza pubblica, e sulla cui effettiva cantierabilità nelle attuali condizioni economiche permane più di un dubbio, per usare un eufemismo, come anche l'attuale Governo sta cominciando lentamente a comprendere. Quindi, di 6 miliardi di euro ne mancano ancora 4,7. In Calabria e Campania l'Alta capacità Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria è stata inserita nel contratto di programma RFI 2007-2011, aggiornato al 2008. Sono previsti in questo caso il quadruplicamento della Salerno-Battipaglia, costo vita 1,8 miliardi di euro, interamente da finanziare, il potenziamento tecnologico della Battipaglia-Reggio Calabria, la variante Ogliastro-Sapri (con un costo vita di 3,2 miliardi di euro, anche questi interamente da finanziare). I due interventi complessivamente, com'è logico, hanno un costo complessivo di 5 miliardi di euro, interamente da reperire. In Puglia e Campania, e veniamo appunto alla questione oggetto della precedente mozione, l'Alta velocità‑Alta capacità Napoli-Bari, con un costo vita, come è stato ricordato, di 5 miliardi di euro, ha una copertura di poco meno di 1,5 miliardi di euro: mancano quindi 3,5 miliardi Il quadro che ho testé rappresentato, pertanto, solo per le opere prioritarie che ho elencato e che sono necessarie alla realizzazione dei progetti TEN è caratterizzato da un costo pari a poco meno di 24 miliardi di euro (23,7 per la precisione), con risorse effettivamente disponibili ad oggi stanziate, colleghi della maggioranza, pari soltanto a 4,5 miliardi euro, poco più di un sesto; va detto anche che se aggiungessimo la nuova linea ad Alta velocità Battipaglia-Reggio Calabria, che costa 18 miliardi di euro, tale cifra già lieviterebbe a 42 miliardi. Se poi aggiungessimo ancora le opere che non fanno parte dei corridoi paneuropei, elencati peraltro puntigliosamente nella nostra mozione - non a caso e che rivestono un'importanza strategica per il Mezzogiorno, fra l'altro inseriti nel piano delle infrastrutture strategiche (tra cui si trova, per ricordarlo, la statale ionica con un costo vita di 15 miliardi di euro, il nuovo collegamento Palermo-Catania e altre opere), il costo salirebbe a quota 67 miliardi di euro, peraltro già ricompresi nel piano per le infrastrutture strategiche del Governo. Al momento, le risorse effettivamente stanziate disponibili ammontano a circa 8 miliardi di euro pari, colleghi, neppure ad un ottavo del fabbisogno complessivo. Questo è l'effettivo stato dell'arte, non altro.

e sulla conclusione dei lavori entro il 2013, in quanto interamente finanziata, della tratta Salerno-Reggio Calabria, sono affermazioni di una tale inattendibilità da commentarsi da sole. sole. Riteniamo che al Parlamento sia richiesto di fare chiarezza e di sgombrare il terreno dagli equivoci. Noi, con questa mozione, abbiamo inteso richiamare il Governo e la maggioranza alle proprie responsabilità, al netto dei proclami e delle politiche degli annunci, che sono forse anche efficaci sul piano della comunicazione e dell'illusorio consenso, ma che lasciano il Paese drammaticamente immobile nelle sue condizioni, un Paese che rischia così di non cogliere l'opportunità di una sfida per l'innovazione di cui l'infrastrutturazione per il Sud costituisce non solo il terreno di intervento più nobile ed alto, ma anche la principale occasione di sviluppo per l'altra metà del Paese. finestra"). Colleghi, è presente in tribuna una delegazione di docenti e studenti dell'Istituto di istruzione superiore "Don Giovanni Colletto" di Corleone. A loro va il saluto dell'Assemblea.

che il Governo ed il Parlamento intendono incentivare per lo sviluppo del sistema dei trasporti nel Mezzogiorno d'Italia. Tutto ciò si articola in un momento di particolare difficoltà economica del Paese, difficoltà nota, sulla quale ci siamo a lungo confrontati, che determina anche politiche di bilancio restrittive con particolare riferimento

Nel sistema del trasporto riferito al Mezzogiorno d'Italia il ruolo delle Ferrovie dello Stato è sempre stato centrale nonostante le difficoltà derivanti dall'assenza di investimenti consistenti per la manutenzione straordinaria e l'implementazione della rete ferroviaria, con particolare riferimento alle Regioni meridionali.

realizzazione del ponte sullo Stretto, che è considerato uno strumento non di collegamento fisico tra la Regione siciliana ed il resto d'Italia, ma attraverso cui realizzare il sistema dell'Alta velocità da Napoli a Palermo. La La realizzazione del ponte sullo Stretto diventa l'anello di congiunzione e di conclusione del Corridoio Berlino-Palermo e dunque lo strumento attraverso cui si ammoderna l'intera rete ferroviaria del Mezzogiorno d'Italia garantendo anche da Napoli

Il ponte sullo Stretto non ha una copertura finanziaria integrale, ma parziale, posto che il resto dell'opera dovrebbe essere finanziato con il concorso di privati, tenuto conto di quali sono le condizioni economiche in cui

la possibilità di portare avanti politiche di investimento in questo settore nel Mezzogiorno d'Italia, che è legittimo il lavoro che Ferrovie dello Stato sta facendo la parola "lavoro" in termini esclusivamente eufemistici perché vi sarebbe tanto da dire su Ferrovie dello Stato e sul suo ruolo in questo Paese rassegnarci ad una conclusione negativa dei ragionamenti che in questa sede il Parlamento, nelle sue diverse articolazioni di maggioranza ed opposizione, sta tentando di fare, in uno spirito costruttivo che parte anche dall'iniziativa del collega Gallo. A ciò vorrei aggiungere un'altra considerazione, poiché la seconda grande direttrice delle politiche di investimento nel sistema infrastrutturale del Mezzogiorno è data dalla realizzazione e dall'ammodernamento

come l'ammodernamento della rete e il conferimento di pari condizioni di competizione economica a diverse aree territoriali, non fanno parte del patrimonio politico di questo o quello schieramento, devono far parte del cosiddetto senso dello Stato. Infatti, uno Stato esiste se tutti i territori sono tra di loro messi nelle condizioni di poter competere ad armi pari. Quando, viceversa

sono impiegate in maniera diversa e prevalentemente al di fuori delle finalità istituzionali, mancano poi le risorse per

risorse. Ci troviamo di fronte ad una condizione di fatto rispetto alla quale nessuno, indipendentemente dal partito di appartenenza, può restare inerte

sarebbero pari a poco più di 116 milioni di euro, con una riduzione di circa 134 milioni di euro rispetto a quanto erogato nel 2008.

al settore del trasporto merci e che consisterebbe in una riduzione di circa 56 milioni di euro. Se a ciò associamo quanto Ferrovie-RFI ha comunicato in termini di contrazione delle risorse rispetto alle politiche di ammodernamento, di manutenzione e di resa in efficienza della rete, su cui opera il trasporto su rotaia, e se poi a questo aggiungiamo i dati che riguardano il taglio e la contrazione delle risorse, sia con riferimento agli investimenti infrastrutturali, sia con riguardo ad un'altra voce importantissima del capitolo relativo al trasporto (cioè il trasporto locale e regionale, in relazione al quale anche è operata una sorta di riduzione), ci rendiamo conto che chi paga le conseguenze

sull'onda dei grandi progetti di lunghissimo periodo, si vede sottrarre quotidianamente risorse in favore di altre aree del nostro Paese. Non me ne vogliate, colleghi della Lega, ma riteniamo che sia una provocazione aver presentato oggi questa vostra mozione, quando tutti i Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, a cominciare dal principale Gruppo di maggioranza (il Popolo della Libertà), hanno voluto concentrare la loro attenzione sull'atteggiamento colpevole di Ferrovie dello Stato (poi bisognerà vedere se si tratta del Governo, cioè del concedente o del concessionario). In ogni caso, mentre si registra un disagio e una difficoltà, sia con riferimento ai progetti che riguardano l'Alta capacità (Napoli, Bari e più in generale la Puglia), sia con riferimento alle opere infrastrutturali e agli investimenti sulla rete ferroviaria nel Mezzogiorno, voi presentate invece una mozione, per carità giustissima, ma che come direbbe qualcuno «non ci azzecca» e sul piano politico e istituzionale va considerata solo una provocazione egoistica che non fa onore al dibattito politico che stiamo svolgendo sul tema, che è uno solo e riguarda gli investimenti che si vogliono fare e che questo Parlamento vuole che il Governo faccia nel Mezzogiorno d'Italia. C'è poi un altro caso nel caso, che riguarda la cosiddetta area dello Stretto,

del servizio, a tal punto che i passeggeri scendono a Villa San Giovanni e proseguono per nave il percorso per raggiungere la Sicilia. Ma ci rendiamo conto, vi rendete conto, che questa è una politica miope e folle? che, mentre l'area degli investimenti nei prossimi anni è concentrata nei Paesi mediterranei del Nord Africa, nella cosiddetta area di libero scambio, l'Italia si presenta a questa competizione globale su quei mercati con una rete ferroviaria che fa così dire «rame da tutte le parti» (visto che viene rubato!), con un'infrastruttura su gomma che non esiste perché cantierata e sarà bloccata ancora chissà per quanti anni e con autostrade del mare che non esistono perché siamo in attesa di capire come il progetto di privatizzazione della Tirrenia riuscirà a sortire quegli effetti taumaturgici che trent'anni di gestione pubblica non hanno prodotto. Questo è il punto politico rispetto al quale, sia la mozione del collega Gallo, che le altre, sono

e rimodulare le priorità per garantire al Mezzogiorno una rete infrastrutturale che gli consenta di produrre ed esportare a condizioni paritarie rispetto alle altre aree del Paese. Se volete fare questo, siamo pronti a farlo insieme a voi, altrimenti assumetevi la responsabilità davanti agli elettori anche su questo tema sotto scopa della Lega che vi porta la mozione per l'opera pubblica del Nord che, ripeto, è solo una provocazione politica di pessimo gusto. Non fate gesti di dissenso con la testa, perché purtroppo è così, colleghi;

per ragionare attorno al tema dei trasporti e dei collegamenti del Mezzogiorno, quindi dell'intero Paese, dell'Italia. Il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che un sistema di mobilità pubblica efficiente un sistema di mobilità pubblica efficiente costituisce un obiettivo strategico per la costruzione di politiche volte a promuovere sviluppo sostenibile e migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nell'ottica e nel rispetto degli accordi del protocollo di Kyoto e del programma di riduzione di gas dannosi dell'Unione europea. Vorrei fare alcune considerazioni di fondo che riguardano il tema centrale, cioè la modernizzazione del Paese e in particolare della regione del Mezzogiorno. mi rifaccio ad una riflessione che abbiamo fatto in 8a Commissione proprio con le audizioni, cari colleghi Filippi e Gallo, e Gallo, degli assessori regionali delle varie Regioni del Mezzogiorno, che ci hanno dato uno spaccato terribile. Quindi, fare oggi una riflessione attorno a questi temi significa assumerci fortemente la responsabilità dei collegamenti del Sud; quando dico del Sud o del Centro-Sud, dico del Paese Italia. In questo ci differenziamo fortemente da una visione leghista egoistica, di parte, che dimostra ancora una volta che è un partito non nazionale ma che si rivolge soprattutto all'area forte del del Nord. Cosa vuol dire la dorsale del Centro-Sud? Vuol dire ragionare attorno ad una situazione di degrado ormai intollerabile che per certi aspetti rappresenta un calvario anche per tutti i nostri fratelli italiani del Centro-Sud. Parliamo del Lazio: la tratta ferroviaria Roma-Pescara è ormai inadeguata ed obsoleta

Parliamo della Sicilia: storicamente le Ferrovie dello Stato non hanno mai concretamente avviato un programma di ammodernamento della rete nella Regione; si parla di 1.444 chilometri

Questo è un dato che evidentemente fa capire a coloro che sono già intervenuti che senso ha fare il ponte sullo Stretto di Messina. Parliamo della Calabria, che risulta avere una flotta di treni attivi ormai vetusta, che i collegamenti non si riescono più a realizzare. È una situazione critica, certamente imputabile al progressivo abbandono del sistema ferroviario calabrese da parte di Trenitalia SpA. Il trasporto ferroviario della Regione Basilicata è divenuto talmente precario che non si trovano a volte neanche i treni, che vengono soppressi oppure dotati di carrozze sudice e cadenti. Hanno soppresso anche l'Eurostar Taranto-Potenza-Roma. Cosa dire della Regione Puglia che deve sopportare la sostituzione di treni veloci come l'ETR500 delle linee Lecce-Bari-Roma e Taranto-Bari-Milano con locomotori e carrozze vetuste dove ormai si viaggia in maniera penosa? Ma possiamo andare avanti. Allora, secondo Allora, secondo noi, il tema da porre oggi fortemente all'attenzione del Parlamento, del nostro Senato, ma in particolare del Governo, è quello di ripristinare i finanziamenti per l'Alta velocità che riguardano la tratta Napoli-Bari, già stanziati dal Governo Prodi. Il costo complessivo che si ritiene necessario per un rilancio effettivo è di circa 5 miliardi di euro, di cui circa 1,5 risultano finanziati

Il fatto positivo da rilevare, invece, è che il decreto-legge n. 185 del 2008 ha istituito un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato con una dotazione di 960 milioni di euro per il 2009 e una autorizzazione di spesa per 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

chiede di porre in essere davvero ogni atto di competenza del Governo che sia finalizzato a ridurre i disagi dei lavoratori pendolari che pagano sempre i sacrifici per primi, promuovendo in tempi celeri tutti gli atti normativi necessari a scongiurare il rischio della marginalità dei territori, affidando la programmazione dei servizi alle intese tra le Regioni interessate; a reperire adeguate risorse a favore delle Regioni del Mezzogiorno, finalizzate all'acquisto di nuovi treni per pendolari per il servizio pubblico locale, per il rinnovo dei contratti di servizio e per gli investimenti necessari a garantire la sicurezza ed il rinnovamento del parco mezzi; ad accertare l'effettiva rispondenza del servizio di trasporto ferroviario nelle Regioni del Mezzogiorno a quelli che dovrebbero essere gli standard moderni rispondenti ai requisiti di sicurezza, efficienza e qualità; a porre in essere ogni atto di sua competenza volto a garantire i necessari interventi di infrastrutturazione per il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci nel Mezzogiorno; a confermare le scelte assunte con il DPEF 2008-2011 e il relativo allegato infrastrutture proprio per la realizzazione della tratta Napoli-Bari, garantendone il completamento in tempi certi; a porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato a realizzare l'estensione della rete Alta capacità ed Alta velocità nel Mezzogiorno da Napoli verso Salerno, Battipaglia, Reggio Calabria fino alla Sicilia;

a vigilare affinché il gruppo Ferrovie dello Stato non serva in maniera difforme il territorio nazionale e assicuri il riequilibrio dei servizi a favore di quelle fasce di utenza che, non solo sono tagliate fuori dall'Alta velocità, ma anche dai treni veloci. Concludo dicendo che non c'è Italia senza Mezzogiorno e non c'è Mezzogiorno senza Italia. Questo è l'impegno che chiediamo al Governo, se è vero che è un Governo nazionale di tutto il Paese.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, gentili colleghi, ho ascoltato i senatori che mi hanno preceduto e desidero tranquillizzare tutti: nessun egoismo da parte del Gruppo Lega Nord con la presentazione di questa mozione, come affermato dal collega De Toni, nessuna provocazione, come ha detto il collega D'Alia e, tanto meno, nessuna contrapposizione con la mozione presentata dal collega Gallo,

si inserisce in maniera assolutamente fondamentale nel progetto di modernizzazione di questo Paese. Una macchina non può funzionare se non funzionano tutte le sue componenti. Questo Paese non può andare avanti, non può rinascere, se si lavora sempre a pezzettini, a compartimenti stagni, a macchia di leopardo. Quello che abbiamo voluto fare con la nostra mozione è evidenziare questa capacità di interconnessione. Il sistema ferroviario italiano ad Alta velocità/Alta capacità si sviluppa, lo ricordo, per più di 900 chilometri, attraverso il territorio di sei Regioni e di oltre 150 Comuni. Comuni. Geograficamente è strutturato secondo una grande T che parte da Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno per poi proseguire verso Benevento, Bari e Lecce e, dall'altra parte, unisce Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia e Trieste. Queste nuove linee sono state progettate con lo scopo ben preciso di consentire un traffico promiscuo, quindi sia di passeggeri che di merci.

Quindi, le caratteristiche progettuali funzionali delle nuove linee veloci sono state definite in modo da rendere possibile la circolazione, in condizioni di massima sicurezza, di un numero di treni quasi doppio rispetto quello attuale.

Padova-Mestre e la Milano-Treviglio, che erano dei veri e propri colli di bottiglia, a questo punto c'è una urgenza fondamentale rappresentata dalla tratta Treviglio-Brescia-Verona-Padova. La realizzazione di questa linea ha un duplice obiettivo: da un lato fornire collegamenti veloci su lunghe distanze e, dall'altro, alleggerire la rete ordinaria. È quello che chiediamo al Governo e sono sicuro di poter uscire dall'Aula

Ciò consentirebbe a tutto il Paese di essere inserito nel sistema ferroviario della direttrice del Sud Europa. Se questo è solo l'interesse del Nord, qualcuno me lo deve spiegare. A che cosa possono servire

della Lega Nord, presentando questa mozione, sia assolutamente in tema e quindi non generi nessuna contrapposizione con la mozione presentata da tanti illustri colleghi, dal senatore Gallo, come non c'è nessuna provocazione e nessun egoismo da parte nostra. Stiamo lavorando tutti insieme, spalla a spalla, nell'interesse di questo Paese, per prepararci ad affrontare le sfide che dovrà affrontare questo Paese se vorrà rinascere.

Signor Presidente, in una terra, la Sicilia che com'è noto è un fortino elettorale per il Popolo della Libertà e per l'onorevole Berlusconi, vengono prelevate, nascoste, cancellate le risorse necessarie a superare la grave fragilità del sistema dei trasporti. I provvedimenti anticrisi varati dal Governo prevedono un utilizzo delle risorse, i cosiddetti FAS, che sono divenuti il bancomat di questo Governo. Il piano di riparto attribuisce alla Sicilia il 24 per cento delle risorse disponibili; questa quota prevista per il piano di riqualificazione del parco rotabile, pari ad oltre 110 milioni di euro, sommata ai 25 milioni messi a disposizione dalla Regione, avrebbe consentito di aggiornare il parco rotabile ferroviario per il trasporto regionale. Questo Governo ha scippato i finanziamenti per l'ammodernamento della viabilità secondaria, ha distratto i fondi per le infrastrutture e pretende di utilizzare i fondi strutturali europei per finanziare gli ammortizzatori sociali nel Nord del Paese. L'Italia è una, ma la Sicilia ed il Meridione continuano a pagare un prezzo altissimo: la colpa sta anche nel giustificazionismo dei parlamentari siciliani - forse mi sbaglio, farei meglio a parlare di asservimento - a danno dei siciliani che rappresentano. Siamo stanchi di sentire per motivi elettorali il Presidente della Regione siciliana, l'onorevole Lombardo, ritenere poco generoso verso l'isola questo Governo. Siamo stanchi del gioco delle tre carte, tra assessore al bilancio della Regione, onorevole Cimino, il sottosegretario, onorevole, Micciché e il ministro Fitto. Avete portato i pullman dalla Sicilia per manifestare per il ponte, ma perché non lo avete fatto per le ferrovie siciliane? Va bene il ponte, ma vi rendete conto che collegherà due deserti? Siamo ancora senza il doppio binario tra Palermo e Messina, fino a poco tempo fa il treno da Palermo ad Agrigento impiegava cinque ore, a Cammarata si bloccava per danni ai binari, i passeggeri trasferiti in corriera alla stazione successiva e con un altro treno via, felici, verso la città dei templi. Non è un film di Tornatore, ambientato ai primi del '900, non è scritto in un testo di Pirandello: è l'oggi. Venga l'onorevole Berlusconi, con il cappello da bigliettaio e con la paletta da capotreno, parli con i pochi passeggeri si accorgerà di quanti treni Minuetto non sono arrivati e non arriveranno in Sicilia; venga a Palermo: scoprirà che i lavori per una metropolitana inaugurata durante il Governo di centrosinistra, dopo l'avvio, sono stati bloccati da questo Governo. Venga Berlusconi a prendere il trenino per l'aeroporto di Palermo: accolto in pompa magna a Punta Raisi, troverà ad accoglierlo l'amministratore delegato della GESAP in un aeroporto declassato, con meno passeggeri, con *slot* non coperti, con un indotto in crisi. L'amministratore delegato, che ha un compenso molto superiore a quello di un parlamentare, gli ricorderà che con il Governo Prodi aveva comprato due pagine a colori con i soldi pubblici di due giornali per pubblicare l'interrogazione di parlamentari di Forza Italia per rivendicare una certificazione colpita dai ritardi della burocrazia. Dopo il declassamento causato dalla CAI, invece, il silenzio preoccupante in un aeroporto che ha tante professionalità che vanno rispettate, un aeroporto voluto lì da logiche clientelari e gestito da un amministratore delegato che è il primo dei non eletti in questo Senato della Repubblica; logiche clientelari e mafiose in un aeroporto con un nome che qualcuno vuole ancora cambiare, un aeroporto che porta il nome di Falcone e Borsellino per ricordare che in quella terra, ancora oggi, giorno dopo giorno, dobbiamo combattere per affermare la legalità, per utilizzare le adeguate risorse necessarie a far decollare l'economia libera, per far uscire la Sicilia dai *gap* che la fanno vivere ancora in una non risolta questione meridionale. Queste ed altre motivazioni mi hanno spinto a sottoscrivere la mozione di cui è prima firmataria la senatrice Finocchiaro. Chiedo anche ai colleghi

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il tema che solleviamo con la nostra mozione rappresenta la cartina di tornasole per verificare come il Governo e la sua maggioranza intendano affrontare in primo luogo l'emergenza della crisi economica che il Paese sta attraversando e, conseguentemente, quali strategie abbiano davvero intenzione di perseguire per consentire al Paese di uscirne in maniera positiva e proiettato verso una prospettiva di crescita e modernizzazione del sistema economico e sociale nazionale. L'infrastrutturazione logistica e, in particolare, quella ferroviaria costituisce uno dei nodi più rilevanti da affrontare per rendere reale l'obiettivo dell'Italia, piattaforma logistica nel Mediterraneo per l'intera Europa, evitando ancora una volta, dietro a miopie e provinciali litigi, di perdere il treno, come si suol dire, verso il futuro del nostro Paese. Perdere il treno significa perdere finanziamenti, collocazioni negli snodi programmatori sovranazionali, affievolire, qualora ce ne fosse bisogno, il nostro prestigio nelle sedi internazionali dove, soprattutto sul versante delle infrastrutture, si decidono i destini delle economiche continentali La nostra mozione è un richiamo alle responsabilità del Governo e del Parlamento perché, partendo dalla priorità dell'infrastrutturazione ferroviaria al Sud, si dia concretezza e coerenza al completamento di quella del Centro Nord, collegando tra loro quel sistema di corridoi transeuropei che manca, per mettere in relazione i mercati delle economie mature con quelli in piena espansione e con quelli in via di sviluppo. Al cuore del nostro ragionamento c'è il sistema Paese, ma non in termini assistenziali; siamo infatti consapevoli di quali siano le priorità e, di conseguenza, le gradualità, perché si imbocchi finalmente la strada di una politica infrastrutturale in grado di dare non solo nel breve, ma per le prossime generazioni, un sistema più moderno ed in grado di affrontare le sfide della crescita e della competitività in uno scenario non solo nazionale ma almeno europeo. L'Europa, come soggetto unitario, deve garantire a tutti i suoi cittadini e a tutte le sue imprese la massima mobilità interna ed esterna e per fare ciò ha deciso di inserire come priorità nella sua agenda lo sviluppo di un efficiente sistema integrato dei trasporti all'interno del quale il trasporto ferroviario dovrà ricoprire un ruolo centrale. Su 30 progetti prioritari, ben 17 riguardano il trasporto ferroviario, con un'estensione totale di 106.000 chilometri, di cui 32.000 ad Alta velocità, con un dimensionamento superiore rispetto a quello previsto per il sistema stradale, indicato in 96.000 chilometri. Il completamento e, soprattutto, il finanziamento delle infrastrutture strategiche per il trasporto ferroviario costituisce una sfida chiave non solo per l'Europa, ma accomuna soprattutto i singoli Stati membri, che dovranno congiuntamente trovare le risorse adeguate per realizzare questo progetto ambizioso ed indispensabile. Infrastrutture e reti ferroviarie sono altresì mirate a sostenere un mercato competitivo, efficiente ed integrato, dal quale non possiamo e non dobbiamo tenere fuori una parte considerevole del nostro territorio nazionale, che invece può rappresentare una grande opportunità di crescita per l'intero sistema. Si sostiene spesso che il Mezzogiorno sia il problema dell'Italia e da un certo punto di vista non c'è dubbio: se per assurdo il Mezzogiorno facesse parte della Spagna e non dell'Italia il reddito italiano sarebbe più alto. si potrebbe sostenere anche il contrario, ossia che il problema del Mezzogiorno è che si trova in Italia; se per assurdo facesse parte della Spagna, il suo reddito crescerebbe più velocemente. Il problema dello sviluppo regionale in Italia, delle disparità territoriali, del Mezzogiorno, oggi più che mai non può che essere interpretato tenendo conto del quadro nazionale, il quadro di un Paese con difficoltà strutturali, a lungo mitigate dal suo grande dinamismo, ma ormai, da diversi anni, messe a nudo da cattivi da risultati economici. L'una cosa non può che andare assieme all'altra. Non si può immaginare un soddisfacente sviluppo delle Regioni italiane più deboli senza una significativa trasformazione e ripresa complessiva di tutto il Paese. Non si può immaginare una ripresa di tutto il Paese senza una forte crescita delle sue Regioni più deboli. Negli ultimi anni la crescita dell'Italia è stata assai inferiore a quella del resto d'Europa e del mondo e l'andamento è simile in tutte le Regioni. Dal 2003 il Nord va un po' (ma solo un po') meno peggio del Sud, grazie soprattutto al forte aumento dell'occupazione straniera. L'economia del Sud soffre degli stessi mali di quella nazionale, ed in forma più accentuata, e capirne le ragioni significa comunque comprendere anche le difficoltà dell'intera economia italiana. È per questo che la mozione del Popolo della Libertà è del tutto inadeguata ad indicare al Governo un impegno concreto che renda coerenti gli annunci e le reiterate promesse di interventi epocali ai quali non fanno seguito né un euro di finanziamento, né l'accelerazione degli *iter* di realizzazione, né atti concreti, ma solo interventi di tagli e riduzioni degli stanziamenti che vengono dirottati su altri interventi che non stanno producendo alcun effetto. La mozione del Popolo della Libertà è debole, attenta a non far emergere le contraddizioni della maggioranza rispetto ai contenuti della mozione presentata dalla Lega che, invece, usando strumentalmente il tema delle infrastrutture ferroviarie nel Sud, chiede che le risorse siano prioritariamente usate per l'avvio si tratta solo dell'avvio - della progettazione di tratte ferroviarie tra Brescia e Padova; una priorità, si badi bene, che è anche nostra, ma non possiamo

funzione dell'evento dell'Expo, vengano poi utilizzati in senso contrario allo sviluppo che dobbiamo avere nel Mezzogiorno. È per questo che con la nostra mozione chiediamo che si dica qui ed ora se la leva dello sviluppo infrastrutturale è una delle opzioni strategiche che si intende utilizzare per ridare forza e slancio al Paese, se questa strategia è rivolta verso la modernizzazione e la crescita qualitativa del nostro Paese, non contrapponendo ma collegando in modo virtuoso tutto il nostro territorio, da Nord a Sud, nell'interesse di tutti e per il bene della nostra collettività. La realizzazione di un sistema infrastrutturale che faccia dell'Italia la piattaforma logistica del Mediterraneo non è materia di slogan, convegni o *spot*; è tema dell'oggi. E se questo Governo, invece che far prevalere al suo interno i ricatti reciproci, saprà guardare alla sua doverosa missione nazionale, potrà trovare nella nostra mozione le idee e le proposte utili per affrontare non solo l'emergenza della crisi attuale ma una prospettiva di lungo respiro che sia per il bene di tutto il nostro Paese. *(Applausi

sembra sempre senza fine e senza tempo. Si fa fatica a pensare che nel 2009 si debba chiedere per la qualità della vita dei cittadini, in particolare del Sud, un intervento strutturale per ammodernare reti stradali e ferroviarie. È un lamento antico, si potrebbe dire, se non fosse, come ben sanno anche i colleghi Gallo e Mura, che abbiamo ascoltato in Commissione lavori pubblici del Senato esponenti di tutte le Regioni hanno rappresentato con tutta evidenza la diversità delle condizioni fra Nord e Sud, la diversità delle problematiche e la diversità delle richieste. Io mi voglio soffermare brevemente solo sui casi della Salerno-Reggio Calabria e del ponte sullo

al ponte di Messina si sono dette e scritte molte cose, di alcune delle quali ha riferito il collega D'Alia, al quale chiedo di apporre la mia firma Mi sembra improprio invocare sempre quest'opera come se fosse la soluzione di tutte le difficoltà. Non c'è dubbio - e non ce lo dobbiamo nascondere - che il ponte susciti una grande suggestione nelle popolazioni interessate ed è di tutta evidenza che se fosse realizzato costituirebbe un elemento di attrazione di investimenti ed un possibile polo turistico. Ma non c'è dubbio neanche sul fatto che il tema non può riguardare il collegamento tra le due sponde di Sicilia e Calabria. Per far quello basterebbe un buon sistema di traghetti veloci che in venti minuti trasporti dall'altra parte. Il tema invece riguarda, come più volte si dice propriamente, il collegamento con il Paese, con l'Europa, con l'Europa, che oggi è a velocità molto diverse; riguarda il rafforzamento degli investimenti e l'eliminazione delle disuguaglianze. Per questo motivo, ritengo, non ci può essere un prima e un dopo. Bisogna finanziare e definire le infrastrutture stradali e ferroviarie e contemporaneamente portare avanti, se volete, il progetto del ponte sullo Guardando al Sud del Paese non come un problema ma come una risorsa e assicurando a tutti i cittadini d'Italia pari condizioni di qualità della vita, eliminando le differenze, valorizzando la circolazione delle merci e delle persone che in questa società plurale rappresentano, da sole, un veicolo di civiltà e di sviluppo. Noi siamo consapevoli - lo scriveva un grande scrittore siciliano, Francesco Lanza - che siamo stati per troppo tempo abituati a discutere «all'ora del vizio», a crogiolarci sulle nostre presunte virtù e a lamentarci delle ingiustizie. E ci rendiamo conto che dobbiamo guardare avanti. Per questo è indispensabile sostenere una condizione di uguaglianza, perché chiediamo che mai più ci si dica che viene dato a titolo di carità ciò che invece è certamente dovuto a titolo di giustizia. Va bene l'Alta velocità e l'Alta capacità e ci piace che i nostri colleghi chiedano, come hanno fatto i senatori Gallo e Mura, interventi per altri territori. Il problema è spiegarlo in Sicilia, dove è un eufemismo persino dire che esistono le ferrovie. Nel frattempo, riterremmo serio almeno approvare la nostra mozione. *(Applausi

Presidenti delle Regioni Campania e Puglia, il progetto preliminare. Quindi, siamo già in una fase avanzata. Sempre per la verità, devo dare atto e ringraziare il Governo del presidente Berlusconi, il ministro Matteoli e il sottosegretario Castelli per essersi adoperati a che fosse quest'opera, già partita nel 2001, ma che già apparteneva alla programmazione della Regione Campania, quando chi vi parla aveva la responsabilità di assessore regionale ai trasporti, per avviare questo avvicinamento del Mezzogiorno d'Italia alla grande infrastruttura. Credo che già qualche altro collega abbia parlato di questo argomento volendo sottolineare un aspetto: noi del Mezzogiorno d'Italia non vogliamo dire alcunché; reclamiamo soltanto i nostri diritti.

il collegamento ferroviario Napoli-Benevento-Bari-Lecce, che mette al centro la Valle Caudina e il nodo cruciale di Benevento, così come era già accaduto sin dall'epoca dei romani, è semplicemente una una infrastruttura che serve per collegare meglio questa piattaforma naturale, che è il Sud dell'Italia, che estende le proprie propaggini a ridosso del Medio Oriente e dei Paesi emergenti. È il naturale collegamento Est-Ovest del Corridoio 1, Berlino-Palermo, con la continuazione a Bari per Varna e quindi per questo mondo emergente del Medio Oriente che servirà assolutamente non già soltanto a collegare le popolazioni locali ma a creare ipotesi di sviluppo. Su questo punto dobbiamo essere attenti. Presenterò un'ulteriore interrogazione per conoscere l'andamento dei lavori circa la realizzazione

situazione in cui ci troviamo, cioè quella dell'elaborazione del progetto preliminare, debba essere assolutamente velocizzata. Certo, abbiamo come obiettivo finale il 2020, ma stiamo

possibile realizzare. La Regione Campania ha messo a disposizione dei fondi per l'elaborazione del progetto, abbiamo già delle disponibilità, pari a ben 708 milioni di euro

del collegamento con la stazione dell'Alta velocità (che io, da assessore regionale vorrei chiamare Stazione Campania) e quindi del collegamento con l'Alta velocità che proviene da Milano e passa per Torino, Bologna, Firenze, Roma,

quello che da Benevento ci porta ad Apice è già realizzato come raddoppio, dobbiamo andare avanti e fare la Bari-Orsara. Certo, si prevede di realizzare una galleria di ben 28 chilometri compiere uno sforzo economico incredibile (tutta l'opera costerà ben 6 milioni di euro), ma, come ha detto bene il ministro Matteoli, nel suo intervento a Benevento la settimana scorsa,

di avviare tutte le procedure e consentire che questa opera possa finalmente partire con la realizzazione della Variante di Acerra ed il raddoppio della Benevento-Napoli attraverso la Valle Caudina. In merito, vorrei fare un rimprovero forte, determinato e convinto agli amici della sinistra, soprattutto al presidente Bassolino della Regione Campania, quando

mio intervento e ringraziando l'Aula per l'attenzione che ha posto alla discussione di questo argomento, vorrei dire che sono completamente d'accordo con i colleghi intervenuti prima di me che

per svilupparsi e non costituire un appesantimento per il Paese ma una risorsa. La Napoli-Benevento-Bari, con la propaggine fino a Lecce, certamente raggiunge questo obiettivo, perché, come abbiamo già detto, mette in collegamento il Corridoio 1 con il Corridoio 8 e, siccome le nostre linee ferroviarie sono fatte con il sistema bimodale, cioè trasporto merci e trasporto passeggeri, certamente con questa avremo creato le condizioni per lo sviluppo di questa area territoriale. Però c'è bisogno di velocizzare, c'è bisogno di creare le condizioni affinché per davvero dal preliminare si passi al definitivo e per davvero si avviino i lavori.

un Paese che ha bisogno di essere infrastrutturato secondo alcune linee strategiche che il Governo aveva

da noi fortunatamente non sta ancora accadendo, ma ciò non ci deve certo far dimenticare che il momento attuale è molto grave. Il Governo si è interrogato rispetto a due esigenze fondamentali: la prima era cercare di tenere a posto i conti pubblici.

Abbiamo compiuto anche un'altra scelta, definendo come priorità anticongiunturale l'intervento nel campo delle infrastrutture. Ricordo - è uno studio che non proviene dal Governo, ma da Confindustria - che ogni miliardo che riusciamo a spendere nelle infrastrutture di trasporto

il Mezzogiorno in particolare, ma non soltanto. Consentitemi di fornirvi un dato, colleghi: in rapporto agli abitanti, la Provincia che ha meno strade in assoluto in Italia - guarda caso - è quella da cui io provengo, Lecco.

Come dicevo prima, è necessario destinare il maggior numero di finanziamenti al settore delle infrastrutture. Quindi, abbiamo fatto una cernita, attraverso la nostra struttura di missione, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture che ricadono sotto la legge obiettivo,

Non voglio qui fare polemica, non mi sembra il caso, ma mi fa piacere che anche dai banchi dell'opposizione, che è stata al Governo fino a poco tempo fa,

attraverso un'operazione forse anche discutibile - e che è stata discussa - di ripristinare la questione dei *general contractor*, che di fatto avevano bloccato tutte le opere relative alla TAV.

fa parte di quella grande croce Nord-Sud-Est-Ovest di cui si parlava prima. Abbiamo poi cercato di liberare una serie di fondi dei privati,

Dopo il lavoro fatto al Ministero, in cui abbiamo individuato le opere immediatamente cantierabili, il CIPE le ha deliberate, quindi è un passaggio anche di natura politico-amministrativa estremamente importante.

e anche il ponte sullo Stretto di Messina. In un'ottica federalista, credo sia giusto che siano le classi dirigenti locali a stabilire le priorità, una volta che sono state destinate e distribuite le risorse. mozioni) dei 7.300 milioni di fondi FAS è certo, è sicuro, perché lo prevede la legge (direi che diventa ultroneo che lo riaffermi una mozione, ma

cento dei 7.300 milioni di fondi FAS. Il grande progetto che ha messo in atto il Governo vale 16.600 milioni, a cui sono da aggiungere altri 1.200 milioni,

cento verrà utilizzato nel Mezzogiorno: questo vuole la legge, questo vuole l'Europa e quindi non c'è il minimo dubbio. In proposito devo tranquillizzare assolutamente tutta l'Assemblea.

i volumi di traffico del Nord consentono finanze di progetto che stanno in piedi; al Sud questo ancora non accade. Francamente non so se augurarvelo o meno, colleghi del Mezzogiorno, perché significa densità di popolazione che

sulle cosiddette opere calde al Nord abbiamo grandi possibilità sotto questo punto di vista, al Sud ne abbiamo meno; ce ne sono due che stiamo valutando e su questo chiedo alle classi dirigenti del Sud di fare un grande sforzo. Credo che sia giunto il momento in tutto il Paese - qui ho sentito molte volte appellarsi all'unità del Paese - che anche sulle autostrade si faccia in modo che tutti siano chiamati a dare un contributo per il loro utilizzo. Allora, sulla Salerno-Reggio Calabria, quando sarà completata (e sarà completata), ritengo che sia giusto chiamare gli utilizzatori a pagare un pedaggio, come sia giusto farlo sul Grande raccordo anulare con un sistema - lo dico per tranquillizzare il sindaco Alemanno - che non farà pagare i romani ma farà pagare i fruitori; lo stiamo studiando e si può fare: penso sia giusto, così come pagano a Napoli e a Milano, anche per coloro i quali transitano sul Grande raccordo anulare.

ricordo che la prima grande opera, appunto la Milano-Bergamo-Brescia, sta già partendo ed aprirà i cantieri quest'anno; sarà un'opera a costo zero per lo Stato; partiranno che sarà un'opera largamente finanziata dai privati; proseguirà la Salerno-Reggio Calabria, nonostante il gravissimo problema della criminalità organizzata che spesso impedisce ai cantieri di lavorare. Questo è un problema che evidentemente esula dalla responsabilità del Ministero delle infrastrutture, ma è un problema reale ed è uno dei motivi fondamentali per cui spesso i lavori vanno a rilento sul quale credo che tutti insieme dovremmo fare una profonda meditazione. All'interno di questo quadro, credo che possiamo dare un parere sulle varie mozioni dicendo che il Governo ha fatto un grandissimo sforzo per accogliere tutti gli impegni perché lo ritengo giusto ma anche perché molti di questi impegni o sono già in via di realizzazione o sono già previsti dal Governo.

reale: «gli obiettivi di infrastrutturazione dei piani approvati dal CIPE non sempre coincidono con le esigenze di sviluppo territoriali delle Regioni e degli enti locali». Ricordo che il CIPE non decide, ma prende atto delle decisioni il Ministero assume sempre d'accordo con le Regioni. Infatti, tutto il quadro che ho illustrato, in realtà, si concretizza anche all'interno delle intese generali quadro che vengono stipulate con le Regioni. Per quanto riguarda gli impegni,

Posso accettare una formulazione che dica di utilizzare i fondi FAS previsti dalla delibera CIPE in maniera corrispondente alle finalità previste dalla legge,

Sotto questo punto di vista siamo dunque abbastanza coperti. Spero che non si debba erodere in maniera significativa questa cifra. Credo però che nessuno sarà contrario se contribuiremo anche noi ad aiutare

stanziando 480 milioni di euro all'anno per tre anni per il trasporto locale ferroviario. Ricordo che, proprio a seguito del citato provvedimento, in questi giorni il Governo sta firmando un decreto interministeriale tra Ministero dei trasporti e Ministero dell'economia per la ripartizione dei fondi

il Governo è contrario non perché non condivida ciò che viene detto, ma perché credo si sia capito chiaramente che il Governo sta agendo su tutto il Paese. Avrei detto la stessa cosa se qualcuno mi avesse chiesto qualcosa per il Nord

sul quinto, perché è stata una decisione del Ministero del tesoro sulla quale il Ministero delle infrastrutture non ha nessuna possibilità d'intervento, almeno come impegno immediato. Esprimo parere sull'ottavo, perché non è coerente con il disegno dell'Alta velocità. L'Alta velocità è un sistema pensato per collegare rapidamente, non velocemente: la velocità non è il fine, ma il mezzo; dobbiamo collegare non velocemente, ma rapidamente le parti del Paese: sarebbe un assurdo costruire una serie di stazioni sulla strada dell'Alta velocità che la ridurrebbe all'accelerato di qualche anno fa.

a «vigilare affinché il gruppo Ferrovie dello Stato non serva in maniera difforme il territorio nazionale e assicuri il riequilibrio dei servizi a favore di quelle fasce di utenza

quindi, contiamo di farlo partire rapidissimamente; l'interlocuzione con le Ferrovie dello Stato è continua, forse riusciremo ad iniziare i lavori anche alla fine del 2009 o al massimo per i primi mesi del 2010. si tratta di un'opera fondamentale, che vale anche molto. Credo pertanto di aver dimostrato che il Governo sta agendo veramente a livello globale, cercando di intervenire, nel limite delle risorse che si è riusciti a reperire,

Poiché il Governo ha dato una serie di pareri favorevoli con riferimento ad alcune parti dei dispositivi delle mozioni presentate dai Gruppi parlamentari di opposizione (del Partito Democratico, dell'UDC-SVP-Aut e dell'Italia del Valori), che credo troveranno la convergenza ovviamente anche dei colleghi di maggioranza,

in questo stadio è chiaro che la Presidenza non può fare altro che seguire il Regolamento. Se c'è invece una possibilità di riformulazione comune del testo, questo dipende dai

La Presidenza non ha obiezioni a concedere una sospensione di dieci minuti, a condizione che gli altri Presidenti dei Gruppi esprimano il loro parere favorevole. Diversamente, non avrei altra scelta che andare avanti in base al Regolamento.

i voti che saranno dati dal mio Gruppo, vorrei tornare sulla considerazione che il sottosegretario Castelli faceva all'inizio del suo intervento: la considerazione, cioè, che guardare al sistema delle infrastrutture non può soffrire, nella visione del Ministro delle infrastrutture e del Governo, di una una territorialità che separi in due il Paese e che privilegi il Nord piuttosto che il Sud, ma che è l'intero Paese che va guardato ai fini di un disegno e di una predisposizione di un sistema infrastrutturale finalizzato a servirlo

così enunciata, denunci qualche limite nel senso che può essere ulteriormente sviluppata. Cerco di spiegarmi meglio: è l'impostazione di cui ci ha parlato il senatore Filippi nell'illustrazione della nostra Non è un caso che abbiamo fatto riferimento, per disegnare il quadro delle infrastrutture del Mezzogiorno, ai Corridoi paneuropei 1 e 8. Non c'è dubbio alcuno che, almeno in quella che riteniamo essere

- abbiamo voluto sottolineare che il Mezzogiorno si rappresenta oggi come quell'area del Paese che, in ragione della conformazione geografica dell'Italia, della sua piena appartenenza all'Europa e delle decisioni strategiche europee che condividiamo è un perno essenziale per lo sviluppo del nostro Paese affinché gli investimenti che faremo in infrastrutture non vengano penalizzati dalla crisi ma anzi, al contrario, siano finalizzati allo sviluppo del Paese. Tanto più forte sarà la resistenza del Paese alla crisi e tanto più gli interventi sulle infrastrutture potranno svolgere una funzione anticiclica - ne sono assolutamente convinta - quanto più il quadro di riferimento concettuale al quale ci riferiamo sarà quello che vede il Paese avere una grande area di opportunità, che è esattamente il Mezzogiorno. È quanto ha detto poc'anzi il senatore Papania, con una formula che sentiamo troppe volte

del vivere. Abbiamo alcune aree del Paese sottoutilizzate che, peraltro, hanno una posizione assolutamente strategica nel nuovo panorama geopolitico e geoeconomico del mondo, ed è esattamente il Mezzogiorno d'Italia, che a questo punto diventa, proprio nella crisi, una delle aree sulle quali investire perché appunto la funzione anticiclica degli investimenti, anche infrastrutturali, sia di beneficio all'intero Paese ed insieme sia per il Nord del Paese, che ha come sua immediata prospettazione l'Europa, il tesoro, il baule pieno di monete d'oro al quale attingere una relazione con l'Europa alla quale conferire la posizione strategica del Mezzogiorno, una sua infrastrutturazione finalizzata all'intercettazione dei traffici che agiscono nel Mediterraneo, il suo essere lì, nel Mediterraneo, nel quale tornano a parlare le parole della politica del mondo e non soltanto della politica dei Paesi rivieraschi, ciascuno per sé, preso e considerato. Questo era il senso con il quale abbiamo costruito questa mozione e con la quale ne costruiremo altre, che riguarderanno invece la rete dei porti e degli interporti del Mezzogiorno

votazione della mozione presentata dai colleghi della Lega e della mozione presentata dai colleghi del Popolo della Libertà.

però che quella vostra impostazione soffre di un orizzonte un po' più limitato, che è quello del territorio. Insomma, tanto per capirci, se davvero pensiamo che da questa crisi possiamo uscire con un investimento sulle infrastrutture che funzioni anche da strumento anticiclico, non possiamo pensare questo Paese come un insieme di territori, ma dobbiamo pensarlo come una grande piattaforma unica sul Mediterraneo. E perché questa svolga al massimo le proprie potenzialità occorre che l'infrastrutturazione del Mezzogiorno sia adeguata rispetto alla sfida e soprattutto rispetto all'opportunità che l'oggi ci pone. Considero poi - e per questo vi ho apposto la mia firma - molto importanti le questioni sollevate e gli impegni che si chiede al Governo di assumere nella mozione di cui è primo firmatario il senatore D'Alia, ed annunzio contemporaneamente il voto favorevole del mio Gruppo alla mozione presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori.

che non era sicuramente - ripeto testualmente - una rivendicazione territoriale, né un contributo assistenziale volevo mettere le mani avanti perché non vi fosse in questa Aula la solita discussione tra un Sud piagnone ed un Nord che non concede. Ricadiamo sempre in questo ritornello del Sud che soffre e degli altri che ci fanno soffrire: è ora di smetterla, è ora di cominciare a parlare di infrastrutture reali nel territorio. *(Applausi

quasi come una perdita di tempo. Mi meraviglio anche perché abbiamo avuto tante volte in Commissione momenti di confronto sereno: volete far scadere quasi ad un'elemosina

altri. Credo che il contributo unitario sulla crescita del territorio debba venire dalla maggioranza e dall'opposizione. Quando il territorio realizza un'infrastruttura è una vittoria di tutti e non di qualcuno,

e Salerno non debbano essere collegate. Al tempo stesso, ciò non può neanche rappresentare un limite ad una richiesta legittima, inquadrata in un contesto di piano di trasporti nazionale, già prevista, e che la Campania (una Regione non governata dal centrodestra), ha già dotato di un progetto preliminare.

il nostro impegno in favore del territorio. Non voglio parlare da meridionale, perché ho accettato e ho votato il federalismo. C'è chi nicchia, ma io l'ho votato e ho accettato la sfida. Per me federalismo significa che le Regioni devono fare il loro dovere e lo Stato il suo.

per una mozione che ha una serietà, che muove dall'ancestrale sofferenza meridionale e dall'atavico assistenzialismo da cui ci dobbiamo liberare, ad una voglia di competere paritaria e alla necessità di infrastrutture per una sana competizione. dobbiamo tornare indietro, rivendicando assistenzialismo ed il piccolo favore e la piccola precedenza: non è questa la logica della mozione. Se qualcuno di voi gli ha attribuito questo significato, è fuori dai tempi e deve veramente fare un salto di qualità e aggiornarsi.

Prima di passare alla votazione delle mozioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Questo non si è mai verificato ed è una prassi per tutti noi colleghi di quest'Aula - non per una parte in particolare - assolutamente pericolosa, perché lei non può togliere le schede prima che sia aperta la votazione. Non esiste la documentazione della presenza in corso di dibattito; questa è una prassi assolutamente innovativa, signora Presidente, che credo non possa essere adottata perché costituirebbe un precedente estremamente grave. Onorevole collega, io sottoporrò la questione, come altri Vice Presidenti, al Consiglio di Presidenza, in modo che ci sia una prassi consolidata, rimanendo inteso rimanendo inteso che unico scopo della Presidenza è di avere delle votazioni non contestate successivamente. Troveremo, quindi, in una discussione collettiva, la maniera di agire in modo congruo e univoco.

Passiamo alla votazione

La prego, senatore.

Presidente, è chiaro che avevo chiesto di parlare dopo la votazione. Capisco errori nella conduzione d'Aula, ma dare la parola ad un senatore mentre è in corso una votazione non si era mai visto, quindi la pregherei di fare un uso più accorto dei suoi poteri di Presidente. Detto questo,

al senatore, di cui non ricordo il nome, di smetterla di avere un atteggiamento provocatorio che ostacola i lavori del Senato della Repubblica.

assolutamente scandalosa perché questa mattina abbiamo verificato una parità di voti su una mozione sugli italiani nel mondo ed era evidente che vi erano luci accese senza la corrispondente presenza di senatori. Quindi, francamente non capisco il richiamo del presidente Gasparri né i lamenti del senatore D'Alì

i colleghi della minoranza di allora pretendevano continuamente la presidenza Marini. Pertanto, nel momento in cui hanno vinto con due voti rubati ed uno che lei non ha potuto esprimere, avrei ritenuto più giusto che qualcuno di loro si alzasse chiedendo di presiedere l'Aula stato un gesto per dimostrare che questa maggioranza esiste a tutti gli effetti e non con i numeri rubati dentro l'Aula.